L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

attualmente a diversi stadi di avanzamento e destinati ad aumentare e migliorare la capacità e la funzionalità della rete nella Regione, è da segnalare sulla linea Palermo-Messina il raddoppio della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo-Castelbuono. Il raddoppio di circa 32 chilometri è previsto parte in affiancamento da Fiumetorto a Lascari e parte in variante in galleria da Lascari a Castelbuono (Lascari-Cefalù Ogliastrillo di circa 5,7 chilometri e Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono di circa 12 A Cefalù è prevista la realizzazione della nuova stazione in galleria. Per quanto riguarda lo stato di attuazione, Ferrovie dello Stato riferisce che nel 2005 sono state consegnate le prestazioni al *General Contractor* per la realizzazione degli interventi nella tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo. Dopo lo sviluppo della progettazione esecutiva da parte del *General Contractor*, l'apertura dei cantieri è avvenuta il 13 maggio 2008. L'attivazione della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo è invece programmata per il 2011. Il contratto di programma 2007-2011 (aggiornamento 2008), siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, include il progetto «Raddoppio Palermo-Messina» in tabella A04, «Opere in corso», con un costo complessivo di 1.672 milioni di euro circa. Di questi, 728 milioni di euro sono previsti per il raddoppio della tratta Patti-Messina, compreso il sistema di comando e controllo della circolazione; 414 milioni di euro per la realizzazione della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo e 530 milioni di euro per la realizzazione della tratta Ogliastrillo-Castelbuono, compresa la realizzazione della nuova fermata in galleria di Cefalù. Il raddoppio, per carenze di finanziamenti in termini di cassa, nel citato contratto è previsto da realizzare oltre l'arco di Piano. Per dare impulso a tale tratto di raddoppio, nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 è stato programmato di anticipare la realizzazione dell'opera e quindi di consentire l'affidamento dell'appalto principale entro il 2010.

come avete avuto modo di leggere dalle diverse interrogazioni che sono state presentate in questa legislatura, l'argomento sta a cuore a tanti cittadini e senatori della Repubblica,

su come una Regione d'Italia (quindi mi permetto di dire l'Italia) possa accettare una mancanza di collegamenti e di infrastrutture

circa 60.000 presenze di turisti da tutto il mondo. Quel territorio è ancora carico di passaggi a livello

che non soltanto le amministrazioni locali, ma tutti gli enti potessero servire il territorio per quello che merita, ma poi, all'improvviso, ci siamo visti sottratti i finanziamenti.

sua risposta e devo dire che forse questa volta ha avuto molto più peso l'azione del Governo che non quella delle Ferrovie dello Stato.

si completi un'opera che è essenziale da ogni punto di vista. Non abbiamo il tempo per ricordare per quale motivo ciò sia essenziale, ma va da sé per un Paese

Da questo punto di vista, mi distacco forse dal clima *bipartisan* per affermare che in una simile situazione mi appare del tutto fantasioso e fuori luogo pensare a ponti sullo Stretto senza avere prima adeguato le reti

esistono tratte ferroviarie che collegano l'Adriatico al Tirreno che sono state realizzate dai Borboni. Mi riferisco alla

l'ex sindaco di Cefalù. Voglio ricordare che questa è una tratta molto importante, non una semplice tratta, che è inserita nel collegamento metropolitano tra Cefalù e le Madonie, con Palermo e l'aeroporto di Punta Raisi. Raisi. È rilevante anche dal punto di vista delle infrastrutture per la Sicilia e l'Europa, perché questo stesso segmento ferroviario fa parte integrante ed è pertanto coincidente con il Corridoio transeuropeodell'asse ferroviario con il tracciato del Progetto n. 1 del Trans European Network Transport, stabilito con decisione della Commissione europea n. 884 del 2004, asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna/Messina-Palermo; la linea ferrata che si sviluppa lungo la dorsale tirrenica Palermo-Messina; con il programmato nuovo doppio binario Palermo-Castelbuono-Catania-Messina. Signor Sottosegretario, i lavori dovevano già iniziare,

signor Sottosegretario, prima di dichiararci soddisfatti vogliamo vedere la realizzazione di quest'opera, e in maniera *bipartisan*: